perché è pervenuta da parte del Senato una seconda versione del testo. L'esame in Commissione, la discussione generale e l'esame degli emendamenti sono svolti alla Camera dei deputati su un testo che poi non è stato sottoposto alla votazione finale.

se la versione corretta sia la prima versione che il Senato ha inviato alla Camera dei deputati o, in alternativa, se sia corretta e quale sia il testo che ha votato quest'Assemblea, perché in ogni caso, essendovi due comunicazioni, uno dei due testi era sbagliato, e mi chiedo perché. Il sospetto è che, stralciando la parte riferita agli enti di ricerca, si sia sistemato quel difetto di copertura segnalato dalla Ragioneria, corrispondente a 13 milioni di euro.

questi sono problemi della Camera. A me interesserebbe sapere quale testo noi abbiamo votato, quale sia stato inviato e per quale motivo sia stato inviato da parte del Senato un testo errato alla Camera dei deputati. se lei avesse avuto modo di leggere il Resoconto stenografico del Senato avrebbe avuto già risposta alle sue domande. Si tratta

per quanto sommariamente concordiamo sulla possibilità di avere dei benefici per le imprese che poi possono dare l'occasione ai detenuti scarcerati di lavorare, abbiamo sollevato solo alcune considerazioni

Sicuramente l'aver reintrodotto alla Camera i reati continuativi specifici recidivi non è stato un buon servizio. Non si è poi avuto il coraggio di sopprimere

orde di persone che avevano commesso questo reato, mi sono permesso di andare a visitare le 200 carceri italiane per vedere quante erano le persone che sarebbero uscite. Ebbene, da tutte le mie visite è venuto fuori, confermato, signor Sottosegretario, anche dal Governo, che in carcere per *stalking* non c'è nessuno. Quindi, la Camera, in maniera urgente, ha cambiato un testo varato dal Senato

di razionalità o di pensiero: devono eseguire quello che vogliono i giornali, perché sono loro che dettano legge e che scrivono le sentenze. Ne abbiamo una lapalissiana evidenza

diritto. Cari colleghi, non è vero l'assioma che le sentenze vanno rispettate. Voi rispettereste l'intervento chirurgico di un professionista che sbaglia l'intervento e, invece di togliere un rene, toglie il fegato?

così come i medici, gli ingegneri, gli avvocati: chiunque sbaglia, ovviamente in Italia. Non ci può essere una casta al di sopra di tutto che, in nome e per conto del popolo italiano, fa danni, come quello della malagiustizia, che costano 31 miliardi al popolo italiano

molto semplicemente si applichi il dettato costituzionale. La nostra Costituzione all'articolo 13, quarto comma, recita: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». stabilisce: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». L'articolo 28, primo comma, prevede: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti «In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». Ancora, all'articolo 32, primo comma, si legge: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti», Senza contare poi i dettami dell'Unione europea, caro presidente Manconi: bisogna fare di più con la sua Commissione; bisogna costringere il Governo a fare in modo che i trattamenti disumani non vengano più perpetrati nelle nostre nostre carceri. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali all'articolo 3 statuisce: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Ebbene, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte accolto i ricorsi dei proponenti specialmente per quanto attiene a temi legati all'amministrazione della giustizia, sia per quanto riguarda i termini di durata dei

Già dal 1999, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, con l'adozione della raccomandazione n. (99)22, ha invitato lo Stato italiano ad esortare procuratori e giudici a ricorrere quanto più possibile a misure alternative alla detenzione e a limitare il ricorso alla carcerazione, e questo sia per motivi legati ai diritti che per questioni attinenti meramente all'emergenza carceraria. La suddetta raccomandazione evidenzia - leggo testualmente - che «l'ampliamento del parco penitenziario dovrebbe essere piuttosto una misura eccezionale in quanto, in generale, non è adatta ad offrire

e l'Italia soprattutto, aggiungo - «dovrebbero esaminare l'opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli in modo da evitare che essi richiedano l'applicazione di pene privative della libertà». Concludo, Signor Presidente, dicendo che questo è un passo avanti, è una boccata d'aria, ma il problema bisogna ancora risolverlo. In che modo? Con una riforma della giustizia immediata, da farsi urgentemente, perché ce lo chiede il popolo sovrano, e ovviamente,

di alcune forze di maggioranza. Sarà uno scherzo dovuto alla particolarità di questa fase politica, ma riconosciamo che su questo punto c'è davvero un'inversione di tendenza

Abbiamo ascoltato invece con attenzione il dibattito svolto alla Camera e lo abbiamo considerato positivo, a differenza del giudizio di alcuni colleghi, anche perché pensiamo che il testo tornato qui sia migliore di quello licenziato dal Senato, dato che si avvicina maggiormente a quella che era l'ispirazione di fondo del Governo.

invece che sia stata troppo stringente - fortunatamente, dal nostro punto di vista - la pressione che ci ha fatto la Corte di Strasburgo, la quale attraverso una sentenza pilota

Naturalmente pensiamo che questo sia soltanto un primo passo, che si debba proseguire lungo questa strada e che si debba intervenire in particolare su due leggi

Ho sentito dire in quest'Aula che il sovraffollamento è un elemento atavico di questo Paese, il che naturalmente è vero, perché da molti anni a questa parte in Italia ci confrontiamo con un sistema delle carceri particolarmente degradante. È però altrettanto vero che nel corso degli ultimi dieci anni c'è stata, se possibile, un'ulteriore accelerazione delle condizioni di degrado, ritengo che la «legge manifesto» di tutto quello che è stato sbagliato nel corso di questi anni sia la legge n. 251 del 2005,

soffiando un po' meno sul fuoco provocato dalle fabbriche della paura, il tema della recidiva reiterata e della recidiva specifica.

i detenuti che possono accedere ai benefici e alle misure alternative al carcere incorrono nel delitto molto meno rispetto a coloro che invece debbono espiare la pena all'interno delle galere. Si parla di percentuali che, secondo le statistiche,

quanto più libera possibile dalle considerazioni ideologiche e quanto più legata invece alle condizioni materiali. Vorrei dunque concludere il mio

che probabilmente c'entra poco con la discussione odierna, ma che c'entra moltissimo con la necessità di affrontare fino in fondo le questioni aperte che riguardano la giustizia italiana.

Uno spacciatore tunisino, che si chiamava Bohli Kaies, la notte del 5 giugno è stato sottoposto allo stato di fermo da una pattuglia dei carabinieri in Liguria, nel Comune

alle difficoltà e ai guai giudiziari di persone che non sono né spacciatori e nemmeno tunisine. E siccome io penso che lo Stato debba tutelare in maniera sacra (se posso usare

Quante persone usciranno dal carcere con questo decreto? In che misura? Come si farà a quantificare? Nessuno lo sa. Cos'è che cambia, però? Cos'è che è importante? È importante che i nostri cittadini vedano

È vero, sono degli esseri umani quelli che devono entrare in carcere. Lo sappiamo che sono esseri umani, ma in un sistema vero di diritto, uno deve sapere che se commette un reato va in galera e paga. dal Gruppo LN-Aut)*. Deve essere concessa la possibilità di redimersi, la possibilità di rivedersi e la possibilità di essere rieducati, ma se noi andiamo a parlare dei recidivi

che parla di mettere in libertà persone che hanno commesso reati. Non è questa la maniera di affrontare i problemi. Facciamo strutture penitenziarie nuove, facciamo quello che è necessario fare. Questo commissario, cosa fa? Dobbiamo sapere a che livello è il piano carceri. Dobbiamo veramente risolvere il problema, e non continuare a procrastinare una situazione che ci porta a questo tipo di soluzioni tampone, che non fanno nient'altro che destabilizzare il cittadino che non riesce più a capire, in primo luogo, cosa facciamo; poi, se esiste un codice penale, che reati ci sono, cosa stai facendo. Una persona fa qualcosa e non sa neanche se è un reato.

trovato dai carabinieri, immediatamente dopo, con un paio di forbici che tentava di scassinare. Questi sono i casi che ci troviamo di fronte.

Ditelo voi a questa gente che cosa deve fare. Non dobbiamo creare uno Stato dove uno - che non si dica e non si voglia! - pensa di potersi fare giustizia da sé.

C'è il problema delle vacanze. Ma quale problema delle vacanze? Qua abbiamo un problema di reati, di sicurezza e di certezza della pena!

Non abbiamo bisogno di arbitri. VOCI

rispetto a chi viola le regole della convivenza civile. Da questo punto di vista sentiamo sinceramente di non avere bisogno di lezioni da nessuno, ma crediamo anche necessario che lo Stato di diritto favorisca la creazione di tutte le condizioni, non solo per difendersi dai delitti, ma anche per poterli prevenire e soprattutto impedire in futuro. Certo, nessuno di noi s'illude di cancellare

è direttamente collegata alla visione che abbiamo dello Stato di diritto, dei valori della Costituzione, del nostro essere parte dell'ordinamento democratico.

per l'affermazione di alcuni valori e per il completamento di un processo, avvenuto trent'anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale con l'avvio della legge Gozzini, che dovrà trovare ulteriori miglioramenti e cambiamenti sulla strada della ridefinizione del nostro sistema sanzionatorio e degli strumenti limitativi della libertà personale per rendere la comunità più protetta e tutelata rispetto alla diffusione dei delitti.

per cento. Credo che l'efficacia di un provvedimento come questo non possa essere valutata in sé, per quello che stiamo facendo oggi:

Questo è il modo per dare concretezza al provvedimento che stiamo varando e agli altri provvedimenti che completeranno il quadro generale di riforma di riforma di tutto il sistema dell'esecuzione della pena nel nostro Paese. Questa è la cultura che ci deve ispirare. Questo è il modo per affrontare il problema e queste sono le ragioni per le quali, ad un provvedimento sicuramente parziale

di tante questioni che sono estremamente serie e che certamente, voglio ribadirlo, non possono essere sottoposte né alla comicità né all'ilarità dell'Aula, però c'è uno Stato di diritto che compete allo Stato: le leggi, che lo Stato si dà attraverso i suoi organismi democratici, devono essere rispettate in primo luogo dallo Stato. Stato. Non si può pretendere che i cittadini rispettino le leggi, se poi lo Stato, laddove ha la responsabilità, non rispetta le leggi che autonomamente e liberamente si è dato. È evidente che la situazione nelle carceri non rispetta questi non rispetta questi principi di Stato di diritto. I regolamenti carcerari ci sono e c'è la nostra Costituzione che dice che la pena deve avere una finalità rieducativa. Si, nelle nostre carceri c'è una finalità di tipo pedagogico, ma non rieducativa: le nostre carceri molto spesso sono università della criminalità; si entra in carcere con un'esperienza empirica, magari in alcuni settori soltanto e si esce con la "laurea" molto spesso in altri settori, perché la promiscuità,

pena, ma le convenzioni internazionali, le sentenze dei tribunali internazionali; lo dice, qualche volta, anche qualche nostro l'azione dello Stato per ricreare le condizioni dello Stato di diritto all'interno delle sue istituzioni, quelle più delicate, è un obbligo, non una facoltà; non ci può essere manifestazione folcloristica o altro degli amici e colleghi della Lega che può farci derogare da questo principio. Dobbiamo riportare la legalità nel nostro Paese a tutti i livelli, nella politica, nelle istituzioni e nei corpi dello Stato (mi associo alle considerazioni del collega De Cristofaro: questo fatto accaduto nei giorni scorsi è grave e deve essere verificato nei suoi vari aspetti), e dobbiamo riportare lo Stato di diritto nelle nostri carceri. Due parole di verità sulla questione dell'indulto, perché il luogo comune è una cosa, mentre i dati sono già stati richiamati dal collega Susta. L'indulto ha prodotto beneficio aggiuntivo;

L'indulto ha una funzione deterrente in questo caso, perché se commetti un nuovo reato devi scontare la pena che ti è stata indultata. Questo mi pare che, da un certo punto di vista della deterrenza, abbia un'efficacia dimostrata. Voglio dare atto - in questo senso dissento dal collega De Cristofaro - alla tanto vituperata legge ex Cirielli

che sono riconosciuti nelle statistiche, ha avuto anch'essa un effetto benefico e, quindi, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare; dobbiamo riconsiderare con il massimo dell'oggettività le questioni e i fatti come essi sono. un'ultima considerazione. Credo che dobbiamo smettere di pensare che il carcere possa essere il toccasana di tutti i comportamenti criminali. Lo dico anche rispetto alla problematica di questi giorni: lo Stato di diritto si garantisce, se la pena è certa (non c'è dubbio), se la pena è equilibrata e se siamo in grado di farla applicare con giustizia.

sua conversione, pur mantenendo le perplessità di un'inadeguatezza, che certamente registriamo per alcuni punti. una questione che ho posto con gli emendamenti e che ha trovato accoglimento solo in un ordine del giorno: noi abbiamo il dovere di rassicurare e rasserenare l'opinione pubblica - e in questo sono d'accordo con i colleghi della Lega - ma la risposta non può essere soltanto il carcere. La risposta sono i controlli elettronici che la tecnologia moderna mette a disposizione e le diverse pene che possono essere applicate in alternativa al carcere. Pertanto,

i punti in discussione, i provvedimenti di legge e le analisi dei fenomeni sociali, politici ed economici senza il peso del bagaglio ideologico

diciamolo allora a chi ci sta ascoltando: non stiamo parlando - per fortuna, aggiungo - di un provvedimento di indulto o di amnistia. Non stiamo liberando nessuno, stiamo cercando di calibrare due grandi vergogne, tra le tante che abbiamo in questo Paese: la vergogna di avere un sistema carcerario indegno di un Paese civile, che costringe migliaia di cittadini e non cittadini in condizioni indescrivibili - e riavvertiamo la vergogna del nostro essere italiani ogni volta che verifichiamo, al di là dei provvedimenti sanzionatori dell'Unione europea, le condizioni in cui teniamo la popolazione detenuta - e la vergogna di non essere stati capaci - non noi, scusateci, ma il sistema politico che ha governato negli ultimi decenni - di creare un sistema di amministrazione della giustizia che sia equo, rispettoso, ragionevole e degno di un Paese civile. Se la continua a parlare alla pancia e a sobillare la paura, allora l'aspettiamo al varco, per sapere quali saranno le sue determinazioni quando si parlerà, non già dell'extracomunitario in carcere, ma magari del *leader* di una forza politica i cui destini politici dovranno essere valutati anche dai colleghi della Lega! Diciamo anche, ai colleghi della componente SEL del Gruppo Misto, che, dall'altro lato della campana, continuano a richiamare valori più o meno condivisibili (non voglio qui entrare nel merito), chiudendo però

libero da bagagli ideologici, da interessi da tutelare, da affari che si possono concludere nella compravendita e nella dismissione degli istituti carcerari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Noi siamo liberi! Non siamo così presuntuosi da pensare di essere migliori e perfetti: abbiamo tanto da imparare.

noi ci siamo approcciati al provvedimento in votazione analizzandolo. Vi sono due parti distinte da valutare: una è quella che attiene ai provvedimenti relativi alla popolazione carceraria e quindi alla possibilità della detenzione domiciliare (e non già della libertà nelle strade),

per le preoccupazioni fondate, non già su sospetti o pregiudizi ideologici, ma sulla verifica pragmatica dell'esperienza dei commissari straordinari nel nostro Paese: di un'esperienza fallimentare, dietro alla quale molto spesso si sono nascosti, si nascondono e temiamo si nasconderanno interessi torbidi.

rientrasse in quelle categorie di reati messi in sicurezza, cioè per le quali non fosse possibile la detenzione domiciliare insieme a quello di *stalking*, di cui tanto si è parlato e a cui si è provveduto con lo stratagemma francamente singolare di aumentare la pena (lasciamo stare

pragmatico. Con il nostro voto contrario vogliamo dire ai cittadini ed alla popolazione detenuta che non abbiamo messo alcun ostacolo, anzi abbiamo cercato di favorire

Innanzitutto una premessa: fino ad oggi, in questi tre anni e mezzo, il commissario straordinario non ha creato neanche un posto in più in alcun carcere.

deputati, è stato posto un limite alla possibilità di derogare al codice degli appalti. Questo un poco ci rassicura, ma non abbastanza da giustificare il nostro voto favorevole, perché dietro la possibilità di dismettere le grandi carceri storiche, quelle che insistono nei centri storici di grandi città come Roma, Milano o Catania

immobili carcerari, farà la sua operazione «fiato sul collo». Staremo con il telescopio o con il microscopio a verificare l'assoluta trasparenza di ogni operazione di dismissione del patrimonio immobiliare affinché non possa rappresentare un'operazione di guadagno in favore degli amici o dei soliti amici degli amici,

Credo che questo si possa rivendicare come un risultato di una maggioranza composita (anche con il contributo di una parte della opposizione) e di una corretta dialettica fra i due rami del Parlamento. Un testo, presentato dal Governo per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, è stato significativamente migliorato dal lavoro intenso e proficuo del Parlamento, grazie alle modifiche apportate in sede di conversione sia dalla Camera dei deputati Va innanzitutto ricordato l'innalzamento a cinque anni del limite previsto per la custodia cautelare in carcere (articolo 280, secondo comma del codice di Spesso si cita la sentenza Torreggiani in relazione al sovraffollamento carcerario ed alle condizioni dei detenuti, ma si dimentica di citare le raccomandazioni in essa contenute, specie per quanto riguarda l'applicazione della custodia cautelare e la sua durata, che dovrebbero essere ridotte al minimo, compatibilmente con gli interessi della giustizia. Con questa misura abbiamo pertanto contribuito a conformare la nostra legislazione alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed alla giurisprudenza dei suoi organi di controllo in materia di custodia cautelare. Giova ricordare che il 40 per cento circa dei detenuti nelle carceri italiane è composto da persone sottoposte a custodia cautelare in attesa di giudizio, e dispiace dover constatare che la metà di essi, sarà alla fine dichiarata innocente. Abbiamo perciò contribuito ad ottenere un duplice risultato: è stata data una risposta efficace al problema del sovraffollamento, dando un concreto cenno di riscontro alla decisione della Corte Corte europea dei diritti dell'uomo e, contemporaneamente, si è posto un freno all'abuso che si fa della custodia cautelare, spesso utilizzata come strumento d'indagine. L'aumento della pena per il reato di *stalking*, introdotto dalla Camera dei deputati e confermato dal Senato, aggiunge a tali obiettivi la tutela delle persone vittime di un reato spregevole, come quello delle persecuzioni. In questo senso va l'altra importante modifica apportata dal Senato in sede di prima lettura, che, intervenendo sulla disciplina degli arresti domiciliari, stabilisce che il giudice, nel disporre tali misure, debba valutare l'idoneità del domicilio in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa. Con l'articolo 1 viene data una risposta al fenomeno delle cosiddette porte girevoli: le detrazioni di pena saranno anticipate, in modo da limitare l'ingresso in carcere per brevi periodi di detenzione. Nello specifico, per particolari categorie di condannati (donne in gravidanza, madri di prole di età inferiore a dieci anni, persone in condizioni di salute particolarmente gravi) qualora debbano scontare una pena inferiore a quattro anni, se si trovano in stato di libertà, potranno accedere alla detenzione domiciliare senza necessariamente fare ingresso in carcere. Tuttavia, grazie all'intervento della Commissione giustizia del Senato, tale sospensione dell'ordine di esecuzione della pena non potrà essere disposta per i condannati per delitti di incendio boschivo, furto in abitazione e furto con strappo. L'articolo 3 del decreto legge interviene sull'articolo 73 del Testo unico in materia di stupefacenti, che disciplina la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il testo originario del decreto-legge interveniva per consentire al condannato tossicodipendente di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in prima lettura, il Senato ha introdotto requisiti ulteriori per l'applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità; in particolare, il lavoro di pubblica utilità potrà essere disposto solo con riferimento a un diverso reato commesso per una sola volta, in relazione alla propria condizione, e si dovrà comunque trattare di un reato di modesta entità e non dovrà essere un reato contro la persona. Il Senato ha inserito, inoltre, l'articolo 3-*bis*, per sostenere il reinserimento lavorativo degli ex detenuti. In particolare, il comma 1 interviene sugli sgravi contributivi per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, mentre il comma 2 concede un credito di imposta alle imprese che assumono detenuti,

L'articolo 4 amplia i compiti assegnati al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, che potrà continuare nella sue attività di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, senza tuttavia sottovalutare l'importanza delle piccole strutture carcerarie, il Senato ha aggiunto l'obbligo di una relazione annuale al Parlamento, ed alcuni emendamenti, approvati dalla Camera dei deputati, hanno limitato il potere derogatorio sul codice degli appalti. Come vedete, seppure in maniera sintetica, ho citato alcune delle numerose e più significative modifiche sostanziali e positive introdotte dal Senato nel corso della prima lettura, che in gran parte sono state confermate dalla Camera dei deputati; modifiche che sono in linea e spesso rafforzano lo spirito originario perseguito dal decreto-legge, imposto dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, di un'incisiva azione di deflazione penitenziaria, senza che ciò possa significare la rinuncia alle ineludibili istanze di sicurezza dei cittadini. La sentenza Torreggiani del gennaio 2013 ha condannato lo Stato italiano a causa dell'assenza, nell'ordinamento interno, di efficaci strumenti di tutela dei diritti dei detenuti, in specie sul versante della lesione prodotta dal fenomeno del sovraffollamento. Questo decreto rappresenta una prima risposta urgente: l'obiettivo è favorire la decarcerizzazione degli autori di reati di modesta entità, fermo restando il ricorso al carcere nei confronti dei condannati per reati di particolare gravità. La reale urgenza del problema non può più consentire - lo dico agli amici della Lega e anche al Movimento 5 Stelle - strumentalizzazioni o divisioni ideologiche, o la ricerca del consenso. È necessario dire la verità: non è un indulto mascherato o un'amnistia; è il momento della serietà, della responsabilità, dell'affermazione dei principi previsti dall'articolo 27 della Costituzione e dall'articolo 3 della Convenzione europea Ciò che occorre chiarire con forza, allora, affinché non esistano margini di ambiguità, è che non si tratta di uno sconto di pena: le pene rimangono, così come sono state erogate, restano le condanne, non si scalfisce la certezza della pena; si cambia l'esecuzione della pena in alternativa al carcere, in coerenza con l'obiettivo del recupero sociale e della riabilitazione declinato dalla nostra Costituzione, che corregge in senso moderno e coerente con il suo spirito solidaristico il principio della pena come valore in sé, come retribuzione senza altra ragione se non quella afflittiva. nostro esame è dunque motivato da ragioni che ogni cittadino può apprezzare, perché di buonsenso e di civiltà giuridica. Da questo punto di vista, quindi, questo intervento legislativo non vuol dire arretrare di un centimetro rispetto all'azione di contrasto al crimine, anzi, chi è pericoloso socialmente non potrà avere altra possibilità che questa e le altre leggi consentono. Questo provvedimento rappresenta, come dicevo, una vera e propria misura strutturale, un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, certezza della pena e recupero del condannato; così come integrato e arricchito nell'*iter* parlamentare, sarà capace di incidere sostanzialmente e positivamente sull'ordinamento penitenziario. Ecco il senso del lavoro fatto a più riprese in Commissione, È un primo passo, lo ripeto: è giusto e necessario compierlo. Per affrontare questa situazione ci vogliono misure di emergenza come queste previste in questo momento e interventi di più lungo periodo che stiamo trattando trattando ancora nelle Commissioni. È per questi motivi che annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà a questo testo legislativo, nella convinzione che il cammino per riportare la pena detentiva e le condizioni delle carceri italiane verso una completa e definitiva revisione e riorganizzazione non si ferma qui. Che questo provvedimento rappresenti il primo passo per creare quel clima di condivisione necessario - richiamato dal Capo dello Stato - per affrontare la riforma della giustizia, quella riforma che gli italiani ci chiedono per una giustizia giusta per tutti. *(Applausi

Quello delle carceri è un tema complesso, molto delicato, ed è chiaro che lo strumento del decreto‑legge non si presta bene ad affrontarne la complessità e a trovare soluzioni ampie nonché condivise in Parlamento. Avevamo la necessità, come prevede la nostra Costituzione, di fare presto, perché l'urgenza è ben motivata. È stato più volte anche ribadito in quest'Aula che la Corte di Strasburgo ci ha rimproverati, ma con la sentenza Torreggiani non si è limitata più ad un rimprovero: ci ha imposto indicazioni ben precise.

Il Senato ha migliorato il testo proposto dal Governo. Abbiamo fatto in modo di selezionare meglio i reati da escludere dai benefici: gli incendi boschivi, il furto in appartamento, il furto con strappo. Abbiamo anche avanzato una proposta, discussa con il Governo e approvata qui in Aula, Aula, chiedendo che i recidivi gravi e specifici fossero esclusi dai benefici, e il Senato così ha votato.

Il bicameralismo prevede queste soluzioni. Su altri punti, la Camera ha migliorato il testo del Senato. Per noi era importante non dare segnali sbagliati sul delitto di finanziamento illecito dei partiti:

sia nella fase attuativa sia nella fase di programmazione. Avremo modo di vigilare insieme affinché il commissario non fuoriesca dai binari della legalità nell'accelerare una risposta di cui peraltro abbiamo bisogno. Colleghi, possiamo dire tranquillamente al Paese che abbiamo scelto una via seria e rigorosa: i mafiosi stanno dentro, l'articolo

abbiamo trovato la soluzione che ci aiuta a tenere in piedi la dimensione rieducativa, trattamentale, la possibilità di curarsi meglio, senza cedere ad alcun permissivismo; anche questo punto, riflettere insieme e trovare soluzioni più avanzate. Il carcere non può riprodurre un sistema di discriminazione sociale:

chi è potente, chi è un colletto bianco ha invece mille accorgimenti per evitare il carcere. Dobbiamo evitare questa contraddizione pesante che abbiamo

ecco perché ho apprezzato moltissimo lo spirito di cooperazione e di collaborazione che, in particolare in Commissione giustizia, si è realizzato tra tutti i Gruppi.

ma altre devono rimanere aperte, perché dobbiamo avere un'idea diversa da quella che fino ad ora abbiamo vissuto nel nostro Paese e che non ha dato buoni frutti.

Ci riusciremo? È una sfida aperta e noi del Partito Democratico faremo di tutto perché essa sia vinta. Tale sfida può infatti aiutare il nostro Paese ad uscire dalla crisi, a recuperare fiducia in se credibilità internazionale e a fare in modo che anche su questo argomento il nostro sia un grande Paese e un Paese migliore. Ecco perché annuncio il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento

non c'è libertà di azione e non c'è libertà di svolgere la funzione di senatore. Ho già tollerato (e non ho fatto denuncia

E invito anche la Presidenza ad adottare nei miei confronti i provvedimenti che riterrà opportuni qualora io abbia violato qualcuna delle regole. Sono pronto a

I Regolamenti si cambiano. Io non ho niente in contrario a che le sedute della Giunta siano pubbliche. Però, al momento le regole sono queste. E se noi pieghiamo le regole scritte ad ogni comodo nostro,

parlamentari così recita: «I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'ufficio di segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al segreto per quanto concerne i i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori». Questo è l'articolo 3 del Regolamento.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti. Ha la parola il senatore Crimi per illustrare la richiesta.

Ho dato la parola al senatore Marcucci. Senatore Santangelo, la prego di sedersi.

interessi tutti noi e interessi soprattutto gli italiani. Oggi è quasi impossibile trovare in tutti gli schieramenti politici qualcuno che spenda parole di sostegno all'attuale sistema elettorale. Non è solo, o tanto, il disconoscimento reso pubblico da più anni da parte del padre riconosciuto, almeno fino a ieri, il collega Calderoli, ma è proprio impresa impossibile trovare dichiarazioni, prese di posizione o interventi che vantino i benefici del sistema elettorale introdotto nel 2005. Al contrario, da ogni parte se ne evidenziano i gravi difetti. Eppure, da ormai due legislature tutti i tentativi di modifica della legge sono stati vanificati. Dopo otto anni e tre elezioni è dovuta intervenire la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso di un gruppo di ricorrenti che hanno sollevato dubbi di costituzionalità. La Suprema corte ha messo su carta ciò che ognuno di noi ha verificato nella sua esperienza politica prima e parlamentare dopo, ovvero che il premio di maggioranza al Senato crea un meccanismo irrazionale irrazionale che di fatto contraddice lo scopo che vorrebbe perseguire: assicurare la governabilità. «Il *bonus* diverso per ogni Regione», ha aggiunto la Cassazione, «porta a una sommatoria casuale dei premi regionali

delle cosiddette liste bloccate, sottolineando che, con tale legge, è in gioco la libertà del voto quando all'elettore viene sottratta la facoltà di poter scegliere l'eletto. Vi è quindi da chiedersi - cito ritenersi realmente libero il voto quando all'elettore è sottratta la facoltà di scegliere l'eletto e se possa ritenersi personale un voto che è invece spersonalizzato». Il meccanismo delle liste bloccate è responsabile anche di un altro disastro: la progressiva disaffezione dell'elettorato. Quante volte, in quanti consessi, in quante iniziative anche di partito, siamo stati avvicinati da cittadini, da elettori, da amici che ci hanno detto: se avete già deciso chi deve andare in Parlamento, se non sono io a scegliere con il mio voto, ma il vostro segretario, beh, allora io alle urne non ci vado In pratica, con il porcellum si è scientificamente rescisso il legame vitale e fondamentale, proprio di ogni democrazia rappresentativa, tra il parlamentare e il suo collegio, tra il parlamentare e la sua comunità di riferimento. Prima mi riferivo ai tentativi di modificare il porcellum andati a vuoto nel corso degli anni. Uno degli ultimi, che molti di voi ricorderanno, risale all'autunno scorso, quando il tema centrale del dibattito politico, anche allora, sembrava essere quello della legge elettorale. Alla Commissione affari costituzionali del Senato, anche grazie allo stimolo dell'allora presidente Enzo Bianco, i partiti hanno discusso e litigato molto su come modificare quella attuale. Poi arrivarono dicembre e la crisi di Governo a vanificare qualsiasi ipotesi di modifica. L'anno scorso, venendo meno a quell'impegno di mandare definitivamente in soffitta il porcellum, ci siamo assunti tutti noi, una pesantissima responsabilità, una responsabilità politica che non chiama in causa tutti nello stesso modo. Non chiama in causa, ad esempio, il collega Roberto Giachetti, che il 5 luglio dello scorso anno cominciò uno sciopero della fame che durò 123 giorni. Abbiamo perso un anno: questa è l'amara verità. Ed un anno e una elezione dopo ci troviamo alle prese con una legge che sarà sancita come incostituzionale e che non ci possiamo davvero più permettere di mantenere in vita. Ci voleva ancora una volta un'iniziativa politica corsara, come la richiesta della procedura d'urgenza avviata alla Camera da Giachetti e al Senato dalla collega De Monte, a cambiare l'ordine delle priorità politiche di questa legislatura. C'è voluta, e ne sono felice, la chiara, netta presa di posizione del Presidente del Consiglio a sgombrare il campo da interessate illazioni, come quelle paventate da alcuni che volevano iscrivere la volontà di cambiare la legge elettorale al tentativo di intralciare o interrompere l'attività dell'Esecutivo. Ha scritto infatti il presidente Letta: «Ottima procedura d'urgenza decisa alla Camera per la legge elettorale. Ora ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Io sono no porcellum». Noi oggi qui stiamo tentando di cambiare questa legge elettorale perché è indegna di un Paese democratico, perché ha alterato i meccanismi della rappresentanza parlamentare, perché ha creato più ingovernabilità, perché ha ulteriormente indebolito la relazione tra eletto ed elettore. Noi oggi qui abbiamo l'obbligo di cambiare urgentemente questa legge elettorale, anche per emendarci delle responsabilità del passato, anche per accogliere, seppure con mesi di ritardo, gli appelli e i moniti del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio. Se allora siamo partiti con la richiesta di procedura d'urgenza, sottoscritta da ben 100 senatori dei vari Gruppi, sulla base di ben sette disegni di legge depositati in questa legislatura che prevedono in varie forme il ripristino del Mattarellum, perché colleghi, abbiamo l'esigenza di rileggere la storia parlamentare e politica degli ultimi decenni attraverso i sistemi elettorali che si sono via via adottati. Una storia che non può che cominciare con la stagione referendaria avviata da Mario Segni all'inizio degli anni Novanta, e soprattutto con quel secondo *referendum* del 18 aprile 1993, data simbolo della politica italiana. Quel giorno gli italiani decisero di cancellare il sistema di elezione del Senato, una scelta che fu interpretata come una svolta in senso maggioritario e antiproporzionale. È il senso di quella svolta che dobbiamo oggi preservare e rafforzare, partendo, ad esempio, dalla chiarezza e dalla governabilità garantita dalla legge elettorale per i Comuni e per i sindaci. Ha questo Parlamento la forza e la capacità di approvare e di condividere un sistema elettorale radicalmente nuovo, nel bene e nell'interesse del Paese? È una domanda alla quale oggi non sappiamo rispondere. Per questo partiamo da ciò che intanto è doveroso fare: abrogare il porcellum partendo dalla strada più facile per raggiungere tale obiettivo, ovvero iscrivere all'ordine del giorno della 1a Commissione e poi dell'Aula i disegni di legge che prevedono il ritorno al Mattarellum. Mi auguro, colleghi senatori, che questa scelta avvenga nel più breve tempo possibile e nel modo più ampio e condiviso. Lo dico senza venature polemiche, ma come presa d'atto di una realtà che si è fatta strada anche nel centrodestra: dobbiamo evitare fino all'ultimo strappi e divisioni sulla materia elettorale. Più ampia sarà la maggioranza che approverà il nuovo sistema e meglio sarà per le istituzioni e per il Paese. In cambio, certo, ci deve essere un patto, che purtroppo è venuto meno anche alla fine della scorsa legislatura: basta melina, basta ritardi strumentali. Dobbiamo evitare che si ripeta la storia del 2005, quando per la prima volta nella storia repubblicana si votò una legge elettorale contro metà del Parlamento per predeterminare un risultato alle elezioni che si svolsero l'anno successivo. Mi sono andato a rileggere i Resoconti parlamentari di otto anni fa, quando, il 13 ottobre 2005, la Camera mandò in soffitta il Mattarellum e approvò il porcellum, che due mesi dopo fu licenziato definitivamente dal Senato. Voglio rendere onore alla lucida previsione di due colleghi che intervennero allora in Aula ed azzeccarono in modo scientifico il futuro che ci è toccato in sorte. Mi riferisco agli onorevoli Ugo Intini e Sergio Mattarella. (socialisti democratici italiani) contraria alla nuova legge: «Si creerà un Parlamento non di eletti, ma di nominati». E come l'esponente socialista, anche il padre della legge che si decise di abrogare, Sergio Mattarella disse: «State cercando di fare in modo che chi governerà dopo di voi debba operare in condizioni meno stabili e più difficili». Oggi, e concludo, superando calcoli di parte e valutazioni interessate, possiamo tutti insieme, cari colleghi, dare una risposta alla fame di democrazia,

Signor Presidente, ho capito che ho la parola. Sto cercando di capire perché si agitano. Sono stato educato così, a rimanere in silenzio quando gli altri si agitano. Ora esercito il mio diritto, visto che mi ha dato la parola. Le leggi elettorali, quando si fanno, hanno degli obiettivi da raggiungere. Quando venne approntata la legge elettorale, di cui ci ha narrato una parte rilevante della storia il senatore Calderoli poche ore fa,

fissare il sistema politico italiano nella normalità europea; consentire tenuta e stabilità dei Governi. Se noi esaminiamo quale di questi tre punti sia stato raggiunto e realizzato nel corso di questi anni, mi pare che nessuno dei tre possa essere considerato raggiunto. La ragione per la quale sottolineiamo e sottoscriviamo le ragioni dell'urgenza della modifica della legge elettorale attuale

libertà che ci consenta, quindi, di scegliere liberamente le mosse di ciascuno di noi. La legge, che ha soprannomi straordinari ed eccelsi, ha raggiunto invece tre obiettivi rovesciati: alcuni di questi figli della situazione politica e sociale italiana, altri legati ad una condizione che questa legge ha peggiorato. Con questa legge elettorale noi abbiamo fatto una cosa che un tempo si faceva rispettando la Costituzione: abbiamo modificato la Carta costituzionale deprivando il Capo dello Stato di poteri infissi nella Costituzione e abolendo di fatto la centralità del Parlamento prevista nella Carta costituzionale. Con la legge elettorale esistente abbiamo aiutato il sistema politico italiano a diventare più dipendente dai partiti personali, in forma bicolore e non soltanto monocolore. Spesso i partiti personali, sono partiti padronali. Abbiamo rovesciato un motto inglese che è stato alla base della democrazia: il motto «senza un partito non un *leader*» l'abbiamo rovesciato in «senza un *leader* non esiste un partito». È il*vulnus* più grave portato alla storia della democrazia occidentale dal secolo scorso. La terza condizione che abbiamo negativamente raggiunto è che non abbiamo aiutato i cittadini italiani a tornare a preoccuparsi e a occuparsi della cosa pubblica.

che ci consenta di fissare un criterio. Poi, quando avremo fissato la cornice del sistema politico-istituzionale futuro, potremo arrivare ad una soluzione definitiva. Questa scelta, illustrata prima dal senatore Marcucci, ne porta dietro altre, ma soprattutto ne porta dietro una, ed è la declinazione dell'articolo 49 della Costituzione esattamente come lo aveva interpretato l'allora onorevole Calamandrei. tratta di una declinazione che manca e che ha aperto nel tempo un *vulnus* privo ancora di cicatrice nella storia istituzionale italiana, perché a partiti esistenti può corrispondere un articolo 49 della Costituzione non declinato e non interpretato, ma a partiti deboli, fragili o inesistenti deve corrispondere per forza un articolo 49 della Costituzione che dia ordine alla struttura e alle tante architravi della democrazia italiana. Questa urgenza ci porta nella condizione di sconfiggere la furbizia di Bertoldo che, come risaputo, non trovavamai un albero al quale farsi impiccare. Oggi l'albero bisogna trovarlo e l'urgenza serve a questo, ma consente anche compagno Briatore di passare finalmente un'estate serena,

Lo facciamo convintamente perché abbiamo anche noi espresso, attraverso la presentazione di un disegno di legge, la necessità di modificare il sistema elettorale in Italia.

che renda più debole dal punto di vista della governabilità il nostro sistema Paese, ma nello stesso tempo non è più tollerabile che la rappresentatività possa essere così annacquata, in queste liste uniche e in questa impossibilità

Non molti giorni fa il Governo ha ottenuto, da un ampio schieramento anche in quest'Aula, il sostegno per affrontare le riforme costituzionali

e continuiamo ad immaginare e a volere, e per questo lo ribadiamo in questo intervento oggi in Senato - che la legge elettorale non possa che essere coerente con l'impostazione delle modifiche istituzionali che vogliamo apportare.

ma non trasformiamo il nostro voto di oggi, il percorso che andremo a realizzare in Commissione e poi in Aula, in un *de profundis* definitivo per le riforme costituzionali che abbiamo già incardinato

non roviniamo ciò che abbiamo già, in maniera veloce e concreta, avviato. Si può realizzare questo lavoro in parallelo, e condivido la posizione del senatore Nencini: intanto mettiamoci in regola dal punto di vista costituzionale e restituiamo un minimo di agibilità

Allora, se oggi affermiamo con convinzione che vi è un'urgenza istituzionale, democratica, dettata dalla Corte costituzionale, di modificare il sistema elettorale

il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ritiene che la legislatura abbia il dovere di fornire al Paese gli strumenti per l'avvio di una stagione in cui le istituzioni siano parte integrante della società. I personalismi e le lotte corpo a corpo degli ultimi giorni

modificare il noto detto nel seguente modo: dichiaro, quindi esisto. Oggi sembra che il certificato di esistenza in vita del politico sia determinato da ciò che riesce a dichiarare o a far riprendere dalle agenzie di stampa. Eppure, vivendo la vita parlamentare, ci accorgiamo che, al di là dei proclami o del breve volgere di gloria di un titolo su un giornale, il Parlamento ha

in omaggio un lavoro che come Gruppo abbiamo svolto. Esso dimostra che non è detto che ad un assetto istituzionale di un certo tipo

allontanamento dei cittadini dalle istituzioni e di disaffezione, legato non soltanto alla cattiva politica ma anche al fatto che la politica non era stata in grado di modificare una legge elettorale che aveva dato vita a Parlamenti di nominati, senza garantire assolutamente - come si

nel sistema democratico del nostro Paese, un distacco forte tra il Parlamento e i cittadini, avrebbe dato vita ad uno strapotere dei segretari di partito e, purtroppo, ahimè, tutto ciò si è verificato.

due pregi; garantiva un meccanismo di scelta da parte dei cittadini, perché il sistema dei collegi fa sì che ci sia un rapporto molto più diretto tra i cittadini e il parlamentare, e tra il parlamentare e il territorio

al riguardo, approfondendo meglio la questione del sistema elettorale. Quello che però a noi preme - ed è questa la questione fondamentale - è che non ci siano più alibi non ci siano più alibi da parte dei partiti e dei Gruppi parlamentari, che non si trovi l'alibi, come ho ascoltato in qualche intervento, di aspettare le riforme costituzionali, ma si proceda senza alcun indugio con la procedura

rinviando le scelte sulle riforme costituzionali, per abrogare il porcellum. Questa sarà la possibilità che noi metteremo in campo, prima del pronunciamento definitivo della Corte, per ricreare, anche se non sarà semplice, cittadini nei confronti delle istituzioni. Spero davvero che questa volta sia il Senato che la Camera facciano sul serio, che ognuno si assuma le proprie responsabilità nel votare oggi la procedura d'urgenza e nell'avviare rapidamente tutti i percorsi nelle Commissioni competenti per abrogare il porcellum. Questo sarà un atto davvero importante, molto più importante

l'esponente del partito socialista intervenire con strali rispetto alla legge. Ieri ho detto che c'erano i nanetti di destra e di sinistra che avevano chiesto l'abbassamento degli sbarramenti; oggi dico chiaramente che il partito socialista fu uno dei richiedenti l'abbassamento degli sbarramenti per cui potesse essere eletto anche il migliore dei perdenti.

ricorda, ma anche in anni passati. Lei ha esordito dicendo che non c'è stato uno che ha espresso una parola di lode per questa legge elettorale. È vero,

perché Rifondazione Comunista non avrebbe dato i suoi voti per il ritorno al Mattarellum. Ma c'erano i voti della Lega, quindi c'era una maggioranza: pertanto, non lo si è voluto fare. Non si abolì il porcellum per tornare al Mattarellum perché Veltroni era convinto che con quella legge avrebbe vinto. Tutto qua, e restò in campo

l'inventore delle liste bloccate sono gli allora DS, oggi PD; siete stati voi a inventare le liste bloccate, voi toscani, perché lo hanno fatto in Toscana il primo esempio di lista bloccata nella storia del nostro Paese. Poi bisogna anche prendere atto che se si vogliono rinnegare completamente le liste bloccate è giusto che non si richieda l'urgenza per un disegno di legge in cui non ricordo se 178 o 173 seggi sono ancora su liste bloccate: se si devono eleggere, si eleggano tutti alla stessa maniera, dai generali ai soldati. Tenere 173 seggi alla Camera solo per i generali, "n' va minga Però cerchiamo di chiarirci le idee rispetto all'*iter* che dovremo seguire. Inizialmente avevo sentito una parte sostenere che le riforme elettorali dovessero essere conseguenti alla riforma costituzionale. È una strada, una linea di pensiero. Qualcuno dice: mettiamo in sicurezza l'attuale legge elettorale anche in vista della valutazione della Corte costituzionale. Qui c'è una incertezza, perché tra i disegni di legge di cui si richiede l'urgenza da una parte ci sono quelli che effettivamente hanno un carattere di transitorietà; ve ne sono almeno due o tre che invece introducono una riforma complessiva a regime che sembra contraddire, mettendo per iscritto il numero dei deputati e dei senatori nella legge, la volontà di ridurre il numero di deputati e senatori. Su questo credo che se la riforma dovesse essere realizzata fare un rinvio a quello che sarà il numero ridotto nella Costituzione, senza congelare una situazione attuale. Ho citato la Corte costituzionale. Ma voi siete così sicuri la Corte costituzionale ammetterà il ricorso e si pronuncerà sullo stesso? Io non ne sono così convinto perché sarebbe la terza volta che la Corte costituzionale, anche se per motivi diversi, esamina questo provvedimento. Si è già espressa due volte per via dei *referendum*, dando un messaggio al Parlamento perché si cambiasse qualche dubbio sul fatto che la Corte costituzionale possa dichiarare incostituzionale una legge che è obbligatoria, perché in qualunque momento potremmo essere chiamati a dovere usare una legge elettorale; sulla possibilità che la dichiari incostituzionale, così come ho dubbi che una sentenza interpretativa così estensiva possa far rivivere il Mattarellum oppure possa introdurre una soglia al di sopra della quale scatti il premio di maggioranza. Non bisogna pensare alla Corte costituzionale né come tagliola né come risolutivo del problema: è la volontà politica che bisogna metterci, ed è quella che chiedo quest'oggi. Ieri, a chiusura del mio intervento, ho detto che è curioso il 31 luglio si esprima la Camera e oggi siamo qui noi a dichiarare l'urgenza, e ho anche sospettato che potesse essere il motivo per un conflitto tra i due Presidenti Camera e Senato per non arrivare ad una soluzione. Ho un suggerimento, e richiamo l'attenzione della presidente Finocchiaro,

per una competizione rispetto ai colleghi della Camera, che qualche volta ci vuole, ma anche perché sono convinto che la Camera che inizia l'esame di una riforma elettorale non possa essere quella che - piaccia o non piaccia - è più figlia del "porcello",

Presidente, colleghi, il Gruppo Scelta Civica voterà a favore della dichiarazione di urgenza. Ricordo che l'attuale Governo (un Esecutivo di emergenza, come sappiamo) ha vincolato - e ha fatto bene ha fatto bene - la propria durata ad un percorso efficace e tempestivo di riordino istituzionale. È importante che, superata questa fase, inizi un percorso nuovo, con elezioni realmente decisive per stabilire chi governa, in grado di realizzare il programma di legislatura sottoposto agli elettori, in un quadro aggiornato ed equilibrato che comprenda nuove garanzie e contropoteri. E ciò non può accadere solo con una riforma elettorale. Ma, come andiamo ripetendo da un sacco di tempo e come abbiamo sostenuto anche nel corso della discussione sulle procedure circa la modifica della Costituzione, c'è l'esigenza pressante di uscire dal porcellum, da quella porcata, per usare una celebre definizione, di cui - abbiamo appreso ieri - è stato vittima il senatore Calderoli. Ognuno la racconta come vuole, ma la vera ragione del porcellum è un'altra. Allora (vi ricordate?) la Casa delle Libertà prendeva più voti nell'arena proporzionale, dove i partiti si presentavano da soli, rispetto all'arena maggioritaria, dove la la coalizione si presentava con candidati comuni. È stato così nelle elezioni del 2001 (la differenza è stata di oltre un milione e mezzo di voti) e nel 1996; per l'allora Ulivo era vero il contrario. Tra le ragioni di questi diversi rendimenti delle coalizioni, c'era il fatto che l'elettorato del centrodestra tendeva a votare i partiti della Casa delle Libertà, ma non sempre i suoi candidati nei collegi. Ecco perché si è voluto modificare la legge elettorale. Naturalmente questo tentativo non aveva niente a che vedere con l'idea di ridurre la frammentazione, di garantire la formazione di coalizioni meno eterogenee, più stabili. Il fatto era molto più semplice: si riteneva di poter guadagnare qualcosa di più nella sfida elettorale e soprattutto di minare la stabilità del Governo successivo. questo è il punto: la vera porcata, mi si passi la celebre definizione, è proprio quella di usare la legge elettorale o le riforme costituzionali come terreno di un possibile incontro, di mediazione tra partiti che sono in conflitto tra loro sul terreno delle politiche concrete,

Oggi come allora, il dibattito parlamentare dovrebbe chiarire proprio questo: se la riforma possa consolidare o indebolire il bipolarismo, se possa incrementare o ridurre la frammentazione del sistema dei partiti e se, soprattutto, essa favorisce o meno la capacità dei Governi di durare e di decidere. Sono queste le domande alle quali dovremo rispondere e che rappresentano i nodi da sciogliere per migliorare effettivamente il funzionamento della nostra democrazia. questo vale anche per l'oggi, perché ci sono dei problemi strutturali e costituzionali che in parecchi fingono di non vedere, come quello di un Governo appeso ai risultati elettorali di due Camere diverse, con i giovani tra i 18 e i 25 anni che votano solo alla Camera dei deputati dell'articolo 58 della Costituzione, il cui comportamento elettorale è per ora molto diverso dal resto della popolazione. Dunque, anche allineando la formula elettorale del Senato a quella della Camera, non è affatto detto che il vincitore risulti lo stesso Quindi, o si toglie il voto di fiducia al Senato o si allineano gli elettorati, facendo votare anche i giovani tra i 18 e i 25 anni al Senato. Senza questo intervento costituzionale resta alto il rischio di nuove elezioni non decisive. Anche la restaurazione del Mattarellum non produrrà risultati così immediati, e non soltanto perché si tratta di ridisegnare e di riscrivere i collegi, ma perché qualsiasi legge che si basi su collegi uninominali - che è la soluzione a mio modo di vedere migliore per il rapporto tra eletti ed elettori - di per sé non produce un sicuro vincitore delle elezioni in presenza di tre schieramenti quasi equivalenti. Più in generale, da circa vent'anni la strada di una razionalizzazione

È vero che questa innovazione è stata incoerente, incentivando contemporaneamente la bipolarizzazione e la frammentazione, e anche regressiva - questo è il caso del porcellum - ma va anche detto che, al netto di questi interventi questi interventi contraddittori, il sistema non è sembrato in grado, anche se fosse stato meglio sollecitato, di configurarsi come una base idonea al funzionamento di una forma di Governo parlamentare efficiente, di una forma di Governo parlamentare efficiente, perché essa richiede una strutturazione, se non proprio bipartitica, almeno bipolare, con coalizioni coese intorno ad un partito guida, la cui *leadership* interna, di partito, ed esterna, di Governo, sia unificata e indiscussa inoltre che il numero dei componenti della coalizione sia limitato. Essa richiede insomma un altro sistema politico. In assenza di questi requisiti di base, le leggi elettorali non possono funzionare come norme di razionalizzazione, o lo possono fare ben poco. poco. Come sappiamo, la vita di questo Parlamento può essere breve e c'è l'esigenza pressante, come dicevo prima, di uscire dal porcellum, specie se si considera che l'ordinanza della di cassazione, che ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, pone il problema politico di individuare soluzioni ponte capaci di sanare i due grandi difetti legislativi indicati: bisogna quindi fare presto.

è più semplice prevedere il superamento *soft* delle lunghe liste bloccate, per cui sarebbe sufficiente la spagnolizzazione delle attuali circoscrizioni ad un livello provinciale o pluriprovinciale. Invece, per quanto riguarda il possibile carattere recessivo del premio di maggioranza, ciò richiede un chiarimento sulle finalità, perché se si persegue l'obiettivo di una democrazia governante, in modo analogo a tutti gli altri livelli di governo, la soluzione più razionale è quella del ballottaggio tra le due liste o le due coalizioni più votate al primo turno, nel caso in cui nessuno

scelta opposta a una democrazia governante, ovvero ripetere con tutta probabilità la strada delle grandi intese obbligate al centro, per un lungo periodo. Lo dico perché il senatore Crimi lo ha esplicitato in una recentissima intervista. Al Movimento 5 Stelle interessa che ci sia meno governabilità possibile per accelerare il crollo del sistema; giova che ci sia più sistema proporzionale possibile per imporre di nuovo le larghe intese in modo che si verifichi la falsa

non va fatta. ad una pratica politica e ad una concezione della politica fondata sulla responsabilità della scelta per il governo del Paese. Scelta Civica sosterrà questo sforzo.

la libertà del voto è stata sempre intesa come divieto di indebiti condizionamenti esterni che incidano sulla determinazione dell'elettore e anche quale necessità di offrire a questi la scelta fra più liste concorrenti e non bloccate. Abbiamo già chiesto, con un'interrogazione scritta, se il Governo intenda costituirsi parte nel giudizio presso la Corte costituzionale e, in caso affermativo, se intenda difendere la legittimità costituzionale della normativa sottoposta all'esame della Corte e se intenda sollecitare la più rapida fissazione dell'udienza di trattazione. A nostro avviso, in quest'Aula ben pochi hanno intenzione di cambiare la legge elettorale. la legge elettorale. Qualche settimana fa, infatti, ci si diceva che la legge elettorale poteva essere oggetto di attenzione da parte dell'Aula parlamentare solo dopo avere messo mano alle riforme costituzionali; bisognava prima cambiare forma di governo e forma di Stato per poi elaborare una legge elettorale coerente con la nuova architettura dello Stato stesso. Adesso, a distanza di pochi giorni, ci fa piacere notare come in tanti convergano verso un obiettivo che ancora 15 giorni fa era sollecitato da ben pochi. Ma qua la coerenza è sempre qualcosa che bisogna trovare con il lanternino. Noi siamo dell'avviso (per quanto magari alcuni di noi studino filosofia)

che ho elaborato anche e soprattutto ascoltando molte riflessioni che, a dire il vero, mi sono piaciute, salvo poi ricordare a me stesso (ancora non ho il morbo di Alzheimer e ho memoria) che proprio chi le produce poi nei fatti adotta comportamenti del tutto dissonanti, per non dire schizofrenici. In molti hanno ragionato sulla libertà dell'elettore: è fondamentale, infatti, in un sistema democratico restituire all'elettore capacità di scelta,

il senatore Calderoli ha indicato chi nel passato - e non soltanto lui - ha condiviso la responsabilità. Quando la libertà dell'elettore è negata da una legge elettorale pensata per ingessare la democrazia e per far sopravvivere la partitocrazia,

allontanamento del cittadino dalla politica. Questo è un risultato che noi, gradualmente, stiamo sempre più percependo, e mi pare che alle ultime elezioni amministrative (e anche su questo vorrei dire qualcosa al collega Marcucci) noi abbiamo, in più casi, ottenuto una percentuale di partecipazione al voto inferiore alla metà degli aventi diritto. Se questa è democrazia, è certamente agli antipodi del nostro modello di democrazia. Questa legge elettorale molti dicono che non l'hanno effettivamente voluta, ma molte battaglie si portano avanti combattendo e non semplicemente dicendo di non volere quello che, effettivamente, non si contrasta (esiste l'omissione di ufficio, l'omissione politica e così via); tutte queste pratiche hanno prodotto una deresponsabilizzazione

ben scarsa consapevolezza, purtroppo, di ciò che spetta loro e di ciò che è loro diritto (oltre a ciò che dovrebbe essere loro dovere) perché,

le responsabilità che invece devono essere di tutti. Ora, noi non vogliamo *leader*, non vogliamo capi, perché, a nostro avviso, in una democrazia siamo tutti *leader* di noi stessi. Il senatore Giovanardi mi sollecita alla memoria un principio che tutti quanti noi sposiamo a parole: *one man, one vote*. Siete voi che avete prodotto, in tante occasioni, e soprattutto in questa,

perché una democrazia sia effettivamente tale, deve essere fondata su un patrimonio di conoscenza che deve essere condiviso. Questo patrimonio di conoscenza lo si può ottenere e costruire quando si lavora su istruzione e cultura, quando non si permette, ad esempio, il conflitto di interessi, su cui non so da quanti decenni noi attendiamo ancora una normativa. È infatti inutile fare la legge elettorale, se poi continua ad esserci un sistema dell'informazione che fa sì che solo alcuni possano farsi sentire e possano raggiungere le libere, in teoria, intelligenze dei singoli, condizionandole. Noi dovremmo ricordarci che la formazione della determinazione, e quindi dell'autodeterminazione del singolo, avviene in funzione della conoscenza. Ma se i materiali su cui si costruisce tutto ciò sono filtrati, sono vagliati e sono selezionati, noi avremo semplicemente una

la legge attualmente in vigore per eleggere sindaci e amministratori locali. Io provengo da un territorio (e sono sempre legato alla alla logica della coerenza), in cui mi ritrovo, nel mio capoluogo di provincia, eletto in Consiglio comunale un consigliere che, eletto nell'UDC, vota e sostiene una maggioranza di centrodestra, mentre, eletto nel Consiglio provinciale in una lista di supporto del Partito Democratico (esattamente Democratici per la Provincia), tranquillamente per una maggioranza di centrosinistra. Siamo arrivati al paradosso per cui sullo stesso atto, quando è chiamata la Provincia a decidere insieme al Comune, lo stesso signore vota con la mano destra quando si trova in Consiglio comunale e con la mano sinistra quando si trova in Consiglio provinciale. Questa è la democrazia che noi rifiutiamo. Questa è la democrazia quantitativa per cui si cerca il consenso a prescindere. Noi reputiamo che il consenso debba essere libero. Ma se deve essere tale, deve essere anche informato. I partiti che ci hanno condotto a questo risultato sono arroccati a difendere queste posizioni. Pochi minuti fa ho parlato con un collega che mi ha detto che non c'è espressamente la volontà poi nei fatti di concordare per un progetto che sia condiviso di razionalità e buonsenso. Noi come Movimento questo chiediamo. Chiediamo razionalità, buon senso giustizia. I cittadini ci chiedono questo. Voi invece avete semplicemente atrofizzato un sistema, permettendo un *vulnus* che era già incardinato nella nostra Costituzione, quello per cui il partito è è tirato fuori dalla possibilità di controllo da parte della legge. Voi avete avallato e legittimato, negli anni, la partitocrazia. Queste sono tesi - torno a ripetere - vecchie come il cucco. Il Paese è in declino. Il Paese - non voglio dire che è in coma - sta vivendo anni bruttissimi perché noi non riusciamo, perché voi non volete cambiare il sistema. Noi siamo qua a rappresentare quella speranza che i cittadini italiani, quelli consapevoli e che sono stati anche capaci

il collega Calderoli in merito alla genesi di quel provvedimento. Non sfuggirà a qualcuno che venivamo da una legge cosiddetta Mattarellum,

In particolare, ricordo che i collegi erano indicati dai partiti come collegi A, B e C: A era quello buono per quella parte politica; B era quello medio; C era quello infimo. Non a caso

Non solo, ma il padre di quella legge - questa volta sì, perché aveva un solo padre, Mattarella - per essere eletto alla Camera, andò in Trentino-Alto Adige a candidarsi.

ma quella che la Nazione in quel momento si merita. Probabilmente quel Parlamento che ha scelto il porcellum meritava quella legge. Infatti, c'eravamo tutti illusi

se questi partiti si attestassero tutti intorno al 25-26 per cento, con la legge vigente un partito che prendesse il 26 per cento, quindi un punto in più degli altri, potrebbe godere di una rappresentanza parlamentare pari al 55 per cento. Questa è l'antidemocraticità del porcellum, che si può verificare. Fino ad oggi la legge non ha mostrato il fianco a una critica così dura, ma sicuramente

Oggi però siamo all'emergenza. Quindi, ci accontenteremo di un dibattito, mi auguro il prima possibile e il più qualificato possibile, al fine di arrivare a una legge elettorale di emergenza - chiamiamola come vogliamo

che si va verso una forma di presidenzialismo o semipresidenzialismo, non può che esserci il doppio turno, cosa che oggi non siamo obbligati a scegliere. Quindi, è necessario che la discussione si faccia il prima possibile.

quale delle due Camere si deve occupare per prima di questo provvedimento. Se fosse il Senato la ringrazieremmo e saremmo pronti ad iniziare nella prima seduta utile l'esame di questo provvedimento.

tutte le proposte, e sulla base di queste ci sarà un libero convincimento. Non sono inoltre d'accordo - e qui anticipo il giudizio sul provvedimento successivo - che ci possa essere l'urgenza per quanto riguarda l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità.

apparato legislativo che, nei casi di ineleggibilità, incandidabilità e decadenza, consente di sapere qual è la scelta che dobbiamo operare. Pertanto il nostro sarà un voto favorevole a tutte le proposte, ivi compresa quella del collega Crimi, che dovremo eventualmente stralciare per la parte relativa alla legge elettorale, mentre il nostro voto sarà convintamente contrario per l'altra parte.

non mi sentirei di sostenere l'urgenza di una legge elettorale a regime. Rispetto invece alla mia richiesta di iscrizione

rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese». Io preferisco che noi informiamo la Camera per raggiungere l'intesa la Camera ci avvisi che ha iniziato. Ricordo ai colleghi che, nella passata legislatura, abilmente il presidente Vizzini dalla prima seduta mise all'ordine del giorno la riforma elettorale e la riforma costituzionale, proprio per impossessarsi di questo argomento. Continuo a ritenere che sia meglio che questo ramo del Parlamento faccia il primo esame e poi lo passi alla Camera con la maggioranza certa, perché, diversamente, una volta iscritto alla Camera, noi ci troveremmo ad approvare un testo bloccato e a non mettere neanche il becco rispetto al ramo del Parlamento che noi

l'8 settembre 2007 ci siamo trovati in tutte le piazze d'Italia in quello che è stato soprannominato il «*V-day».* Quel giorno è nato ciò che oggi ci ha portato qui.

due mandati e il ripristino della preferenza. Erano tre interventi correttivi, in quel momento indispensabili, a nostro avviso, che potevano essere immediatamente resi operativi con la legge vigente,

È bene che la legge elettorale preveda al suo interno anche le cause di incandidabilità ed ineleggibilità. È bene altresì che la legge elettorale abbia stabilità. In questo Paese cambiamo legge elettorale ogni ogni due o tre legislature: quando cambia l'aria, si cambia la legge elettorale per ottenere risultati più vicini a chi

che è stato per sette anni chiuso nei cassetti del Senato, portato in Commissione affari costituzionali e tenuto lì, per due anni,

noi non ci troviamo davanti a un deserto di normativa, ma ci troviamo di fronte ad una normativa che esiste. Quindi, non è materia sulla quale è opportuno dichiarare l'urgenza, come invece sul voto elettorale. Quanto agli argomenti generosamente sostenuti dal collega che mi ha preceduto, sottolineo che essi incontrano il nostro fermissimo dissenso.

tutti quegli annessi e connessi illustrati dal senatore Crimi, allora bisognerebbe avere la dignità di proporre la legge elettorale in Costituzione. voi non l'avete fatto per percorrere quel canale che a voi piace della democrazia diretta, per celebrare quel fatidico 8

nodi oggi vengono interpretati come pesantissimi limiti nel rapporto con la rappresentanza parlamentare, che nel corso degli ultimi anni hanno determinato una vera e propria crisi di legittimità nella percezione delle istituzioni parlamentari: la moralità della rappresentanza parlamentare, la necessità di assicurare un ricambio della stessa rappresentanza, evitando che quella di parlamentare diventi una vera e propria professione (una professione a vita),

e purtroppo lo è già da diverso tempo. La disaffezione dell'elettorato e la sfiducia nella politica e nei politici rappresentano ormai una vera e propria emergenza democratica e probabilmente sono proprio la conseguenza del fatto che per troppi anni questi temi non sono stati affrontati. Noi pensiamo che si possa tranquillamente essere più o meno d'accordo con le ricette proposte da questo

è proprio il motivo per cui esiste il Parlamento, che è esattamente il luogo all'interno del quale i nodi vanno sciolti e le discussioni vanno affrontate. Pensiamo però con la stessa forza che non si può negare l'urgenza assoluta di questa discussione e quindi siamo assolutamente favorevoli,

però vorrei chiarire preventivamente almeno per quanto riguarda noi, per evitare facili e prevedibili polemiche. La decisione di discutere con procedura d'urgenza questo disegno a nostro avviso non può essere collegata, e non deve esserlo, ad un singolo caso, per quanto particolarmente esposto all'attenzione pubblica. nel senso che l'obbligo di affrontare questi temi, a nostro avviso, non dipende dalla loro, peraltro relativa, attinenza a una specifica condanna o ad uno specifico caso di incandidabilità, ma deriva piuttosto dalla necessità urgentissima di ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, tra i rappresentanti e i rappresentati (avrebbe detto un antico maestro) che negli ultimi anni si è spezzato e che il Parlamento, a nostro avviso, ha il dovere di risanare. I cittadini debbono sapere che ai parlamentari si richiede un di più di moralità rispetto ai loro elettori, non un di meno, perché, probabilmente, i privilegi che gli italiani oggi considerano intollerabili risiedono esattamente in questo. E i cittadini debbono poter contare su un rapporto fluido, fondato su un ricambio possibile tra società civile e rappresentanza parlamentare, altrimenti è assolutamente possibile, finanche inevitabile, che si creino meccanismi tipici delle caste. Agli elettori dovrà essere anche restituito (lo faremo anche con la legge elettorale) il potere di scegliere chi li dovrà rappresentare e di non vedersi calare dall'alto i propri rappresentanti. Siccome noi pensiamo che l'esigenza di sanare questi sospesi non è stata determinata da qualche sentenza, non è legata, appunto, ad un singolo caso ma invece esiste da anni e chiama in causa l'intera politica proprio perché ha corroso ed eroso la credibilità del Parlamento e della democrazia, vorremmo che così si interpretasse questo nostro ragionamento. Dobbiamo affrontare queste questioni con coraggio, dobbiamo affrontarle con trasparenza. Probabilmente, anzi, sicuramente avremmo dovuto farlo già da tempo, ed è per questa ragione che ci dichiariamo favorevoli ad adottare ora, con già sulle spalle un inspiegabile ritardo, la procedura d'urgenza.

la procedura d'urgenza per la legge elettorale, ma non voteremo la procedura d'urgenza per questo disegno di legge. Al di là dell'8 settembre 2007, oggi il Movimento 5 Stelle rappresenta il voto di oltre 8 milioni di e incide *pro quota* nel procedimento legislativo. Perché - se tutto è urgente nulla è urgente - non riconosciamo i crismi della urgenza o della opportunità di inserire

avendo, come altri colleghi, partecipato nella precedente legislatura e poi nei mesi o nei semestri scorsi all'approvazione di un disegno serio - sicuramente migliorabile - per un'efficace legge sull'incandidabilità potremmo proporre dei miglioramenti, ma le cronache di questi giorni dimostrano che forse non c'è tutta questa urgenza di un nuovo provvedimento di legge sull'incandidabilità. Finalmente ne abbiamo avuto uno che funziona.

Sulla urgenza della legge sulle incandidabilità parlano le cronache per cui riteniamo, per evitare che siccome tutto diventa urgente poi non ci sono urgenze, che questa richiesta di oggi non abbia e non debba avere nel calendario dei nostri lavori i crismi dell'urgenza.

Pochi istanti fa, all'unanimità, il Senato della Repubblica ha deliberato che l'urgenza è quella della legge elettorale e credo che questa assorba anche ogni altra considerazione circa l'urgenza che viene reclamata dal Movimento 5 Stelle su un'altra proposta di legge, della quale non è il merito ovviamente ad importare, ma il contenuto. rappresentato, per la maggior parte, dal tema delle incompatibilità, come si evince dal titolo della legge, questione sulla quale il Parlamento ha già legiferato in maniera sistematica negli ultimi anni,

È vero che nella proposta del Movimento 5 Stelle c'è una parte dedicata all'introduzione del voto di preferenza. Per quello che vale (ma credo che qualcosa valga dal punto di vista istituzionale), la Presidente della Commissione affari costituzionali dice che quella parte può essere benissimo assorbita nell'esame che faremo del tema della riforma elettorale. Ma il tema dell'incandidabilità è un'altra cosa. Permettetemi anche di spendere qualche parola sulla qualità della discussione che con la dichiarazione di urgenza ci accingiamo a fare. Voglio esprimere qui un pensiero che è assolutamente personale. La mia

legislatura. Noi abbiamo tre obiettivi, com'è stato detto nella discussione odierna: la governabilità del Paese, la scelta degli eletti da parte degli elettori e una maggioranza omogenea e coerente tra Camera e Senato. Questi sono i fini. Intorno ad essi - lo diceva il senatore Bruno poc'anzi - possiamo scegliere tra una quantità di modelli, ma anche rispetto ad una capacità di trovare strumenti che raggiungano questi tre fini, che devono essere considerati le nostre tre stelle polari, ammesso che la metafora possa adoperarsi in questa maniera così imprecisa. Infine, mi permetto di rivolgermi al senatore Morra. Ovviamente quest'Aula serve anche per fare politica, diciamo così, comunque per farsi sentire all'esterno dai propri elettori, per radicare in qualche modo un pezzo della propria identità pubblica. Penso, però, che non possiamo neppure in questo tradire mai la verità. Credo, dunque, di dovermi sottrarre all'accusa che da lei è stata rivolta complessivamente al sistema dei partiti, per cui c'è qualcuno in quest'Aula che non vuole il controllo

del nostro programma, ci teniamo moltissimo e, al di là del fatto che è un testo perfettibile, il fine era esattamente quello. Se i partiti politici rappresentano, secondo la lettera della Costituzione, un pezzo importante della costruzione del sistema democratico italiano

e se, ancora, secondo l'opinione di molti, lo Stato deve limitarsi anche soltanto a mettere a disposizione dei partiti sedi, luoghi e strumentazione, tutto questo vuol dire che, da parte dello Stato, deve

non voglio dire se negli altri partiti si fa o non si fa, o cominciare una disamina dei singoli partiti, ma di certo nel mio partito il segretario viene eletto! Di certo nel mio partito il segretario viene eletto. Anzi, la nostra questione è se debba essere eletto dagli iscritti o da una platea ancora più vasta, con il meccanismo delle primarie. Questo, per dire che la natura di un partito si riconosce da questo, e non è identica nello scenario politico italiano tra tutti i partiti. Era così una volta; non è più così adesso, in un contesto nel quale, invece, si affermano partiti leaderistici che, intorno alla figura del *leader*, si organizzano e si riconoscono e sulla democrazia interna dei quali francamente ciascuno di noi potrebbe anche trovare qualcosa da obiettare. Chiedo scusa all'Aula per aver intrattenuto i colleghi per qualche altro minuto. Come dicevo prima, annuncio il voto sfavorevole del mio Gruppo

è talmente evidente il risultato! Mi dispiace, ma quelle persone che camminavano non erano forse senatori. Li ho visti tutti seduti al

di una ratifica che, come qualche collega magari pensa, si può esaminare in cinque minuti, come spesso accade per le ratifiche. È una ratifica che ha necessità di una discussione approfondita,

fatta salva la necessità di convocazioni per situazioni sopravvenute e urgenti durante il mese di agosto. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 4 settembre alle ore 11, per l'esame di mozioni sui rischi da dissesto idrogeologico, contro la diffusione del gioco d'azzardo, sulla combustione dei rifiuti dei cementifici.

in particolare dei canali della RAI, che hanno causato un disservizio ai cittadini, che tra l'altro pagano regolarmente il canone. Nel corso degli anni, numerose sono state le richieste di intervento da parte delle amministrazioni locali, cui sono succedute le rassicurazioni degli organismi competenti, in prima istanza la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, che non hanno però portato ad una definitiva soluzione dei problemi di ricezione, i quali sono diventati al contrario continui, estenuanti e frustranti. I disturbi al segnale televisivo hanno interessato anche il mio territorio, Biella e l'intera provincia, ma sappiamo che questa è una situazione che vivono altre zone d'Italia, per cui riteniamo che debba esserci un intervento ben più complessivo. Tra i diversi episodi, segnalo quello avvenuto nello scorso dicembre 2012, quando l'assegnazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del canale 23 della banda UHF ad un'emittente locale causò per diversi giorni dei disturbi al segnale RAI, tra la Lombardia e il Piemonte. Questa grave situazione colpisce tutta la popolazione locale, in particolare quella popolazione di *over* 70, che secondo i dati ISTAT, nella nostra zona, supera il 20 Per tali persone l'ascolto del notiziario nazionale e di quello regionale, la cui ricezione è veramente pessima, tutta frammentata, rappresenta un importante veicolo d'informazione, che rischia di venir meno a causa delle difficoltà riscontrate a ricevere il segnale. Quando ci sono poi degli eventi atmosferici di particolare intensità, salta veramente tutto. Visto questo stato di cose, ho deciso di presentare un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico, supportata da moltissimi colleghi del Piemonte, anche di Gruppi diversi dal mio, proprio perché si tratta problema che stanno vivendo moltissime zone d'Italia. Chiediamo quindi di mettere in campo tutte le soluzioni possibili per risolvere in maniera i problemi di ricezione, che ledono la serietà e la credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo, creando disagi ai cittadini non solo piemontesi

quindi portavoce degli idonei, in attesa di assunzione, del concorso per 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, bandito con decreto ministeriale n. 5140 del 2008. Partiamo dal presupposto che è più che mai indispensabile riaffermare l'autonomia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ottimizzandone la funzionalità, attraverso uno stanziamento economico in grado di potenziarne gli organici. Con la disposizione assunta nella *spending review* della riduzione del *turnover* per le assunzioni del personale di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si passa dalla misura del 100 per cento al 20 per cento, nel triennio 2012-2014, e al 50 per cento, incidendo sulla funzionalità e l'operatività del Corpo stesso. Nell'incontro svolto recentemente dalle organizzazioni sindacali con il sottosegretario Bocci sì è riconfermato, con un decreto‑legge,

crea una netta disuguaglianza tra volontari di classe A e volontari di classe B. Le carenze del Corpo nazionale superano le 15.000 unità, secondo gli *standard* europei, quindi riteniamo possibile aprire una fase di assunzione degli idonei del concorso pubblico riducendo così di molto Paradossale appare il fatto che gli aspiranti stabilizzandi - circa 3.000 ancora in graduatoria - devono ancora essere sottoposti ad una prova di selezione motoria e alle visite mediche che ne attestino l'idoneità al servizio, e si dimentica che circa 5.500 unità, appartenenti alla graduatoria del concorso pubblico citato, sono già state selezionate ai massimi livelli e di queste circa 2.000 sono state ritenute idonee al servizio perché sottoposte anche a visita medica. Chiediamo quindi a lei, signor Presidente, di farsi portavoce affinché il Governo si muova in tal senso, per procedere in tempi consoni con le assunzioni del personale del Corpo. Ci sono ragazzi che hanno superato tre prove durissime e una selezione tra 120.000 concorrenti che aspettano di ricevere il posto per cui hanno concorso e per il quale sono risultati idonei. Bisogna che in questo Paese torni a regnare, se mai c'è stata, la meritocrazia.

e anche nelle zone del Campidano irriguo. È una situazione che va evolvendo in modo molto preoccupante. Per fornire solo un dato, Presidente, ogni ettaro di bosco in fiamme ha un valore di circa un milione di euro e gli ettari

Ricorre oggi il cinquantasettesimo anniversario della tragedia di Marcinelle dove, l'8 agosto del 1956, persero la vita di cui 136 connazionali italiani provenienti dall'Abruzzo, dalla Calabria, dalla Lombardia, dal Friuli, dall'Emilia-Romagna, dalla Campania, dalle Marche, dal Molise, dalla Puglia, dalla mia Sicilia, dalla Toscana, dal Trentino e dal Veneto. Vogliamo Vogliamo ricordare il sacrificio di tanti lavoratori italiani che all'estero rendono grande il nostro Paese. Un ricordo e un omaggio a chi, ricercando una vita migliore, ha sofferto lo sfruttamento, la discriminazione e il razzismo. Tutto questo deve essere un monito affinché la vita della persona venga prima di qualsiasi altro interesse. E nel ricordare le nostre vittime vogliamo dire loro grazie per il grande esempio che ci hanno lasciato. Signor Presidente, lei ha fatto gli auguri all'Aula e ai colleghi. Io la ringrazio personalmente e le rivolgo gli auguri, così come ai colleghi, di buone vacanze, ricordando che, contrariamente a quanto i giornali oggi scrivono, questo Parlamento lavora molto più degli altri. Mi permetto di citare qualche dato, anche a conforto dei colleghi, affinché vadano

il 25 luglio e riprenderà i lavori a settembre, in data che deve essere ancora stabilita. I deputati e i senatori francesi hanno un trattamento economico del 50 per cento superiore al nostro. I nostri alacri colleghi tedeschi hanno tenuto l'ultima seduta il 28 giugno

inoltre un trattamento economico che è più del doppio rispetto al nostro, così come i parlamentari europei, che avranno vacanze della stessa durata: dal 4 luglio al 9 settembre. La Camera dei Comuni del Regno Unito ha tenuto l'ultima seduta il 17 luglio e i loro lavori riprenderanno il 30 settembre. Anch'essi godono di un trattamento economico superiore al nostro. Questo anche a informazione dei giornali, che titolano oggi con una sorta di sdegno per le nostre vacanze. Comprendo i direttori di questi giornali che devono dettare faticosamente questi titoli dalle località di vacanza nelle quali si trovano, e speriamo che anche a loro siano utili questi giorni. *(Applausi).*

così come era avvenuto nel periodo passato, a poche iniziative sporadiche di alcuni scellerati, invece quest'anno è riemerso in tutta la sua prepotenza e in tutta la sua importanza.

della fauna; un valore economico, come ha ricordato il senatore Uras, di grande importanza. Oltre a questo, la paura degli incendi tiene lontani tanti turisti dalla Sardegna. io auspico un suo autorevole intervento, come ha fatto il senatore Uras, verso tutte le sedi istituzionali, a cominciare dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e a tutti gli altri che possono intervenire in questa vicenda.

che non si possono processare e condannare tre carabinieri prima ancora che qualcuno abbia scoperto se hanno commesso un qualche reato. Ho fatto presente che, quando Preiti venne fermato davanti a Palazzo Chigi, i carabinieri non gli spararono, ma

detto, e lo sottolineo, che mi rifiuto di considerare torturatori fin da adesso i tre carabinieri, perché non è assolutamente detto che non abbiano fatto il loro dovere. Non gioisco per la morte di una persona. Mi dispiace davvero ma sto dalla parte dei carabinieri e di tutte le forze dell'ordine. Naturalmente so che nei COCER e nei sindacati di polizia la tensione e la preoccupazione sono davvero alle stelle, perché se tutte le volte che si mette a rischio la propria vita per fermare una persona che commette reati si rischia un linciaggio preventivo, chiaro che qualcuno dirà: «Allora andateci voi a fermare la persona che resiste all'arresto». Tutto qui, quindi, non ho gioito di nulla, caro collega, però non me la sento di linciare preventivamente carabinieri e poliziotti quando intervengono per difendere tutti i cittadini.